L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signora Presidente, l'Accordo in ratifica, destinato a sostituire la precedente intesa del 1993 fra l'Italia e la Federazione russa sulla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti, ha portata onnicomprensiva e tende ad istituire una cooperazione nel campo della lotta alla criminalità. La relazione scritta (Atto Senato n.

non contiene previsioni che comportino particolari oneri a carico del bilancio dello Stato. I modesti oneri derivanti dal trattamento di missione del personale di polizia saranno a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.

*(IdV)*. Signora Presidente, cari colleghi, lo spirito con il quale è stata sinora affrontata la discussione della ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa mi sorprende, perché mi è parso troppo generico e limitato. Nel titolo del disegno di legge n. 1302 si leggono le parole e «lotta alla criminalità» e, con il rispetto che come Parlamento abbiamo sempre mostrato verso un accordo internazionale, si tende a dare il generale consenso al provvedimento, senza forse analizzare nel dettaglio il disposto dell'Accordo. Eppure, nel dettaglio degli articoli che compongono l'Accordo sono presenti punti che sfidano lo Stato di diritto ed espongono il nostro Paese ad una collaborazione, senza garanzie, con lo Stato, ben poco democratico, della Russia. Russia. Perdonatemi se tralascerò le considerazioni generali sul fatto che la lotta alla criminalità a livello internazionale è un obiettivo meritorio di essere perseguito con ogni sforzo con l'internazionalizzazione dei mercati, anche l'economia illegale si sia internazionalizzata e, quindi, necessiti di strumenti coordinati fra i vari Paesi per essere Perdonatemi se non concordo su vecchi adagi machiavellici come «il fine giustifica i mezzi» e, quindi, anziché fare un panegirico del giusto fine nella lotta alla criminalità, nell'intervento mi concentrerò sugli sbagliati mezzi, sui mezzi specifici che questo Accordo prevede e sulla disciplina con la quale ciascun articolo li regola. Passo immediatamente all'analisi dei punti in questione. L'Accordo, in sintesi, riguarda la prevenzione e la repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, concernenti la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo, il riciclaggio ed altre tipologie di reato, fra le quali anche i reati informatici. Al fine di condurre tale prevenzione si stabilisce uno scambio di informazioni operative e di carattere giuridico, la ricerca e l'identificazione dei responsabili dei reati indicati, l'assistenza in attività investigative, lo scambio di esperienze e di specialisti, l'addestramento. Nello specifico, l'articolo 1 dell'Accordo regola l'attribuzione delle competenze per l'implementazione dell'Accordo stesso. L'intesa prevede che la cooperazione si effettuerà tramite i rispettivi organi competenti, specificatamente indicati, che potranno essere variati mediante comunicazioni per vie diplomatiche. Quali sono, però, gli organi preposti alla cooperazione?

e di sostanze psicotrope, il Comitato per il monitoraggio finanziario. E per l'Italia? Ne abbiamo discusso anche in Commissione: per l'Italia si occuperà di applicare l'Accordo soltanto il Ministero dell'interno. Colleghi, il fatto che, per ciò che attiene la parte italiana, nell'Accordo manchi la previsione di affidare la competenza ad una pluralità di attori avrà sicuramente due effetti negativi. Il primo è che la mole di lavoro sarà caricata interamente sul solo Ministero dell'interno, il quale, tramite i mezzi materiali ed umani del Dipartimento della pubblica sicurezza, dovrà farvi interamente fronte. Si rischia, sostanzialmente, che nella pratica l'Accordo risulti inefficace per la mancanza di mezzi.

dell'Aula attiene al rischio di una gestione personalistica e senza controlli dell'Accordo. Infatti, far gestire lo scambio di informazioni sensibili e le attività investigative al solo Ministero dell'interno, senza che vadano ad essere interessati pure quelli della giustizia e degli affari esteri, o una Commissione parlamentare, si traduce in una eccessiva personalizzazione e discrezionalità. Sembra che tutta la struttura così verticistica e monocratica vada in contrasto con la nostra architettura istituzionale, basata sulla collegialità, nonché sui freni e i controlli dell'operato dei singoli Ministeri, dei singoli Dipartimenti,

importante. Vorrei porre in luce come nell'Accordo manchino le clausole di rispetto dei diritti fondamentali. Nello specifico, l'articolo 7 stabilisce che il Ministero dell'interno può respingere le richieste russe di informazioni e di cooperazione all'attività investigativa soltanto nel caso in cui queste pongano in pericolo la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Italia. Non viene menzionata la facoltà di negare la collaborazione laddove si vadano a ledere i diritti fondamentali sanciti dalla Carta ONU, dalla Carta CEDU, dal Trattato di Nizza e dai Protocolli OCSE. Non basta un mero riferimento all'impregiudicatezza dei Trattati come si fa all'articolo 9, perché se il Ministero non può rifiutare le richieste che si basano sulla violazione degli stessi, è come se i menzionati Trattati venissero disattesi. Colleghi, riflettete su questi La protezione dei diritti umani è totalmente assente da questo Accordo. È ancora più chiaro tutto ciò se l'articolo 7 L'articolo 2 elenca i reati che sono oggetto di cooperazione fra i due Paesi e, fra i tanti gravi, alla lettera *l)*, si inseriscono anche i reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione. Cari colleghi, non devo neppure menzionare qual è il sistema con il quale la Russia reprime chi si avvale dei mezzi di informazione per dare ai cittadini notizie circa l'operato del Governo; notizie che, se risultano contrarie all'immagine che si vuole costruire della Federazione russa, diventano reati di diffamazione. È tristemente noto l'approccio quasi dittatoriale, al limite del criminale, colleghi. Siamo tutti a conoscenza del trattamento riservato, nel caso più clamoroso, alla giornalista Anna Stepanovna Politkovskaja e poi agli altri operatori del settore, più e meno noti. Non so se ricordate il fatto. *(Richiami del Presidente).* Allora mi chiedo, colleghi: come può l'Italia, una democrazia che garantisce il diritto alla libertà di espressione, sia nell'ordinamento interno, all'articolo 21 della Costituzione, sia nell'adesione a trattati multilaterali, come può l'Italia cooperare scambiando informazioni, nonché ricercando, individuando ed identificando i soggetti sospettati di aver commesso reati, con la Russia che nella medesima materia prevede un sistema penale tanto diverso dal nostro? Non sarebbe stato forse doveroso - e noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo sostenuto in Commissione - inserire in tale Accordo una clausola che vieta di cooperare nel caso in cui il livello di configurazione e punizione di un reato in Russia si discosti dal trattamento penale riservato in Italia per la medesima tipologia di crimine? in caso di urgenza, e in un primo tempo, anche solo verbalmente: Lo stesso vale anche per le risposte. È un atto grave: anche verbalmente si può denunciare un fatto! Ebbene, proprio perché le informazioni e l'assistenza sono finalizzate alla ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, la presenza di documentazione scritta, che specifichi il motivo di dette richieste, è imprescindibile per garantire il diritto di ogni cittadino alle tutele minime in campo giudiziario e Chiedo al Governo di fare una riflessione su quello che sto dicendo, anche al sottosegretario Mantica, sul discorso relativo al «verbalmente», che ritengo grave, almeno per quello che riguarda - continuo a dire - la politica dell'Italia dei Valori, che cerca di far ragionare il Parlamento. Concedere di nuovo una così ampia discrezionalità significa violare lo Stato di diritto.

Di nuovo, questo Accordo appare fumoso, discrezionale, privo di organi di controllo. Se fosse stato concluso con un Paese dell'Unione europea, forse tutte le criticità messe sin qui in luce sarebbero risultate di minore impatto e risolvibili per via interpretativa, in quanto i Paesi europei condividono con l'Italia tradizioni giuridiche, trasparenza e democraticità nella conduzione giuridica. Ma con la Russia le concessioni fatte appaiono, per usare un eufemismo, pericolose e sinistre. Allora, signora Presidente, si deve pensare alla cornice generale, politica ed internazionale nella quale l'Accordo è stato concluso, il 2003, e riflettere su cosa significhino tutte le concessioni che facciamo

Signora Presidente, possiamo dire che stiamo attraversando una stagione abbastanza favorevole per i rapporti internazionali.

Vorrei ricordare e riconoscere anche il merito che ha avuto questo Governo, il Ministro degli affari esteri in particolare, su questo fronte. Abbiamo appena ratificato il Trattato con la Libia, che ha ripristinato i rapporti più distesi possibili con quel Paese, con il quale dobbiamo negoziare in considerazione della grande migrazione che proviene dai Paesi nordafricani magrebini. Abbiamo ratificato il trattato di Prum, che consentirà di avere maggiore sicurezza a livello europeo: penso alla banca dati del DNA del DNA di tutte le persone soggette ad indagini di una certa importanza o pericolosità; alla cooperazione di polizia che potremo attuare; agli sconfinamenti pre-autorizzati (la polizia potrà operare anche al di là dei confini). Sono tutte misure che riteniamo basilari per poter sconfiggere il grande nemico che è sempre più invisibile: una criminalità organizzata a volte meglio degli Stati nazionali.

Cosa significa mantenere rapporti cordiali e distesi con la Federazione russa? Sappiamo cosa sta accadendo, più o meno inconsapevolmente anche la NATO sta compiendo azioni non del tutto funzionali ad una distensione dello scenario europeo. Pensiamo alla pressione che stanno facendo gli americani con le basi missilistiche in prossimità dei confini della Federazione russa,

Ricordo che sono stati gli Stati centrali (Francia, Italia e Germania) ad aver fatto sì che non ci fosse una deriva estremamente pericolosa nel momento in cui metà comunità internazionale si stava per schierare immediatamente a favore della Georgia, non sapendo neanche bene cosa fosse accaduto nel periodo dell'occupazione prima osseta e poi georgiana da parte russa. russa. La Russia si sta affacciando sullo scenario europeo, sta entrando in rapporti commerciali con il mondo occidentale dal quale era sempre stata isolata. Dovremmo far di tutto per non reimpostarla in un nuovo isolamento, che non solo sarebbe improduttivo,

offrire maggiore sicurezza ai nostri cittadini e al nostro Paese. Infatti, va ad incidere su tutta la materia della cooperazione in tema di prevenzione e di repressione dei reati. repressione dei reati. I reati sono quelli che in questo momento più preoccupano tutta la comunità italiana. Coopereremo contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo, contro il traffico illecito tanto di armi quanto di sostanze stupefacenti, contro le importazioni illecite di materiale radioattivo, contro l'immigrazione clandestina, nonché contro la tratta di esseri umani. Lo faremo nell'unico modo possibile in un contesto di rapporti statuali sovrani. Ci sarà quindi uno scambio di informazioni, una cooperazione nelle attività investigative, scambi di esperienze e di

per l'attuazione sul rispettivo territorio. Esso non va a sostituire altri trattati precedenti o futuri sottoscritti reciprocamente dai due Paesi; lascia pertanto

possano normalmente rientrare negli stanziamenti ordinari del bilancio del Ministero dell'interno. Pertanto non necessita nemmeno di una copertura finanziaria *ad hoc*. Riteniamo che il

a causa dell'inversione degli argomenti previsti all'ordine del giorno, il senatore Marcenaro, che avrebbe dovuto prendere la parola a nome del Gruppo del Partito Democratico, mi ha chiesto di sostituirlo

ormai sempre più frequente in sede di discussione di trattati internazionali in Commissione esteri - un dibattito che si è incentrato tanto nel merito dell'Accordo quanto,

con alcuni Paesi, alle volte alleati storici, alle volte alleati più recenti, su una serie di materie, non ultima il controllo della criminalità, che è al centro di questo documento.

riscosso ampio sostegno all'interno della Commissione e l'attiva partecipazione - lo ringraziamo per questo - del Governo nella definizione della sua parte dispositiva. del giorno caratterizza il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico: «Il Senato, in occasione del disegno di legge n. 1302 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, considerato che negli ultimi anni una serie di delitti hanno colpito in Russia persone impegnate nel campo dei diritti civili e in particolare giornalisti e difensori dei diritti umani; che il 7 ottobre 2006 è stata assassinata la giornalista del quotidiano "Novaja Gazeta" Anna Politkovskaja e che i suoi assassini e i loro mandanti non sono stati individuati e puniti; che nella giornata del 19 gennaio 2009 nel centro di Mosca sono stati uccisi l'avvocato Stanislav Markelov, il difensore della famiglia di Elsa Kungaeva, una ragazza cecena seviziata e uccisa dall'ex colonnello Yuri Budanov, e Anastasia Baburova, collaboratrice dello stesso quotidiano di Anna Politkovskaja, a pochi passi dalla Cattedrale di Cristo Salvatore; considerato inoltre che gli assassini hanno potuto agire perché nessuna protezione era stata predisposta per le vittime, nonostante le gravi minacce di cui erano state oggetto; impegna il Governo: nel contesto delle relazioni fra Unione europea e Federazione russa, a manifestare l'auspicio che le autorità russe concludano sollecitamente e positivamente le indagini sui due gravi crimini, identificando i colpevoli e sottoponendoli a giudizio; a chiedere che vengano rafforzate le misure di protezione a favore delle persone che corrono analoghi rischi; a continuare a sollecitare l'Unione europea, sia nel quadro del futuro accordo di partenariato con la Federazione russa, sia nel quadro del dialogo già in essere con quest'ultima in materia di diritti umani, a impegnarsi nella stessa direzione».

semplicemente perché consente di realizzare, anche in Paesi che hanno un ordinamento diverso da quello dell'Unione europea e dei Paesi occidentali,

Vorrei ricordare che la cooperazione tra l'Italia e la Russia si basa su altre convenzioni approvate a livello ONU, e in particolare la Convenzione sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione ONU contro il crimine organizzato del 2000, infine la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 1990. In realtà, attraverso questo quadro normativo di riferimento, che vincola anche la Russia (un Paese con cui l'Italia ha uno stretto rapporto di amicizia e di scambio economico, soprattutto da parte dell'Italia, con un mercato molto interessante per la produzione di alcuni prodotti manifatturieri - in questi Paesi si va delineando ed affermando l'idea che la sovranità, su questo punto, superi l'antico principio per cui sovrano è quel Paese *superiorem non recognoscens*. Anche la Federazione russa, quindi, attraverso questo Accordo (in ordine al quale va sottolineato il merito e l'impegno del ministro Franco Frattini), si assoggetta a queste norme di diritto internazionale e, attraverso il riconoscimento dei diritti e

perseguendo un'omogeneizzazione nelle politiche di sicurezza e soprattutto in quelle di contrasto e cooperazione alla lotta al crimine organizzato ed al terrorismo internazionale. Si deve anche aggiungere che, contrariamente a quanto detto poco fa in alcuni interventi, le richieste verbali che potranno essere formulate agli organi

Signora Presidente, credo che il senatore Divina abbia risposto compiutamente anche alle osservazioni del senatore Pedica, illustrando in dettaglio il contenuto dell'Accordo in esame, che riguarda esclusivamente la lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico di stupefacenti, di armi e ad gravi reati. Ascoltato anche quanto detto dal senatore Perduca per conto del senatore Marcenaro, che dà un giudizio positivo sull'Accordo

signori colleghi, la criminalità organizzata rappresenta senz'altro una delle piaghe più pericolose e difficili da estirpare per la società attuale. Nella forma internazionale, la criminalità organizzata si avvale dei canali di scambio dell'economia illegale e delle difformità tra i vari sistemi nazionali di lotta all'eversione per sfuggire ai controlli.

si sarebbe dovuto compiere attraverso l'armonizzazione dei sistemi penali giudiziari e la formulazione di accordi multilaterali. Questi princìpi sono infatti alla base delle modalità di cooperazione nella lotta alla criminalità che sono state istituite in ambito europeo.

che si interessa alla cooperazione giudiziaria contro le forme gravi di criminalità; l'RGE, la rete giudiziaria europea in materia penale. Si pensi poi nel complesso alla strategia antiterrorismo attuata tramite il controllo delle frontiere con FRONTEX, il mandato di arresto europeo e con le squadre investigative comuni. proprio perché si tratta di tessere una rete volta allo scambio di informazioni sensibili in quanto potenzialmente utilizzabili al fine di punire i responsabili dei reati eventualmente commessi, tale cooperazione, multilaterale o bilaterale che sia, non può avvenire a discapito delle tutele giuridiche che lo Stato italiano deve garantire a ciascun cittadino e a ciascun individuo e nel caso dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa queste tutele giuridiche difettano sensibilmente. Ho sottolineato, in discussione generale, come l'Accordo risulti vago nella determinazione dei meccanismi volti allo scambio di informazioni e alla politica investigativa. Il Gruppo Italia dei Valori anche in Commissione - come manchi una clausola che condizioni la cooperazione del nostro Governo con quello russo al rispetto dei diritti umani. Di qui la nostra sollecitazione al Governo: una sollecitazione - lo abbiamo detto anche ieri

dei diritti umani, che il nostro partito vuole invece sollecitare. Ho sottolineato anche come tutta l'implementazione spetti al solo Ministero dell'interno, con il rischio di una personalizzazione delle relazioni con l'estero, di un sovraccarico

le richieste di cooperazione possano avvenire anche solo per via orale e informale. Per tutti questi motivi, cari colleghi, gestire la materia giudiziaria e di polizia in un modo che è essenzialmente diplomatico, senza alcuna forma di responsabilità verso i cittadini e senza alcun rispetto per le garanzie giurisdizionali poste dal nostro ordinamento, risulta

la prassi degli Stati e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali di condizionare al rispetto dei diritti umani e della democrazia gli accordi, commerciali e non, con Paesi terzi ha conosciuto una grande espansione. Questo principio è denominato, in termini europeistici, clausola di condizionalità. Ma l'Italia con questo accordo del 2003 e con quello libico del 2008 si è sottratta a questa prassi a questa prassi perché, nel firmare gli accordi internazionali, ha preferito perseguire altri interessi, economici o politici, ma sicuramente estranei al bene pubblico: nel caso libico, il guadagno di determinate imprese; nel caso russo, oggi in discussione, i rapporti personali ed intimi tra il nostro Premier ed il presidente Putin. Eppure la politica estera dovrebbe essere condotta dagli Stati, cari colleghi, non dai premier; dovrebbe avvenire tramite canali diplomatici ufficiali, non con telefonate dalla costa Smeralda. Lo ha sottolineato anche il presidente Napolitano nei suoi frequenti moniti in tal senso. Colleghi, che altro dire? Analizziamo e riflettiamo. Le ratifiche vanno sempre votate con senso di responsabilità e noi voteremo favorevolmente alla ratifica. con questo senso di responsabilità vogliamo anche sollecitare il Parlamento ad agire in modo responsabile nelle prossime ratifiche, coinvolgendo il Parlamento,

dal dibattito parlamentare e in Commissione. Chiediamo dunque di riflettere per una politica migliore, per non mettere un bavaglio alle Commissioni

annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord. quali importanti risultati rispetto al passato si stanno raggiungendo e sono stati raggiunti in materia di politica estera da parte di questo Governo.

è l'affermazione e la presa di coscienza che molte forme di criminalità, che minacciano la popolazione e le istituzioni, sono fenomeni sovranazionali, fenomeni sovranazionali, gestiti e organizzati da organizzazioni ramificate in più Paesi e che non possono essere affrontati efficacemente senza un approccio sovranazionale. Questo, colleghi, è dimostrato anche dai pessimi esempi, purtroppo delittuosi, dei recentissimi arresti dei responsabili di alcune violenze ai danni di donne avvenute a Roma, i cui responsabili sono stati in poco tempo individuati ed arrestati, sicuramente grazie alla competenza delle nostre forze dell'ordine, ma

Gli accordi bilaterali e multilaterali contro la criminalità devono costituire principalmente un'assunzione di responsabilità, posto che è innegabile che molti atti criminosi vengono compiuti nel nostro Paese da cittadini non italiani, spesso pregiudicati, che sono già stati incarcerati o ricercati nel loro Paese di origine, o che hanno trovato rifiuto all'Est. Tali accordi devono servire per ottenere quella sinergia di forze, di risorse, di strumenti e di conoscenze atti a massimizzare il contrasto ad azioni criminose, l'opera non meno importante di prevenzione e di pronto arresto dei responsabili e di interruzione delle azioni criminali. Anche questo, Presidente, è quindi un modo per mandare un segnale chiaro ai cittadini, cioè che ogni cosa sarà fatta per consegnare i responsabili dei crimini alla giustizia, per migliorare il benessere e garantire

al contrasto delle tipologie di criminalità che sono svolte in forma organizzata e che investono i settori del terrorismo, del traffico di stupefacenti e di armi, del contrabbando, del riciclaggio, della falsificazione, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli essere umani. Inutile dire con quanta attenzione la Lega Nord intenda vigilare in particolare su queste ultime fattispecie, che rappresentano ormai una piaga internazionale, posto che la tratta di persone è divenuta un'attività di impresa e non possiamo certo continuare a pensare che ogni singolo immigrato decida in solitudine di partire e di venire nel nostro Paese. Al contrario, alle sue spalle ci sono organizzazioni solide e articolate che fanno dell'immigrazione clandestina un vero e proprio *business*. Con questo Accordo, quindi, Italia e Russia si impegnano ad attuare uno scambio di informazioni, la ricerca dei sospettati e la reciproca assistenza investigativa. Ulteriori attività di concerto potranno essere inoltre stabilite di comune accordo, anche con riferimento allo scambio di rappresentanti di collegamento e della determinazione di punti di contatto. è prevista poi l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'identificazione dei colpevoli. Lega Nord voterà quindi decisamente a favore di questo Accordo, auspicando in futuro un più veloce *iter* di ratifica di questo genere di accordi, posto

Presidente, prendo la parola in dissenso dal mio Gruppo, dopo aver espresso nel dibattito generale il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, che confermo anche in questo intervento. Come

purtroppo, ancora una volta (come l'ultimo Trattato firmato con la Libia), faccia economia dell'affermazione del rispetto dei diritti umani, che, in materie come quella della lotta alla criminalità organizzata, credo debba essere ulteriormente affermato. Occorre infatti considerare, per esempio, che un conflitto armato interno alla Federazione russa mi riferisco in particolare a quello in Cecenia, ma ve ne potrebbero essere altri da citare, come quelli in Daghestan e Inguscezia - viene portato avanti come lotta al terrorismo, senza prendere in considerazione alcune delle regole del diritto umanitario internazionale. Il 21 febbraio ricorre, tra l'altro, il 65º anniversario delle deportazioni staliniane del popolo ceceno verso le Repubbliche dell'Asia centrale. Nell'annunciare quindi il voto di astensione della delegazione radicale, comunico che a Milano, dalle ore 14 alle ore 18, si terrà una manifestazione, organizzata dal Partito radicale e dall'associazione Annaviva,

Dal punto di vista contenutistico, questo provvedimento crea le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. stesso. Sul piano concreto, la Convenzione è suscettibile di un forte impatto positivo sulle fiorenti relazioni economiche, commerciali e finanziarie esistenti tra Italia e Stati Uniti, come si evince chiaramente dai dati forniti dalla Banca d'Italia sui reciproci investimenti diretti. conferma e rafforza i rapporti, non solo politici ed economici, ma anche sul piano della cooperazione giudiziaria e di difesa, tra i due Stati, come evidenziato anche dagli altri accordi bilaterali recentemente ratificati dal Parlamento italiano. La ratifica della Convenzione potrà soprattutto rispetto alla crisi economica in corso, che si è tradotta in un rallentamento del volume degli scambi internazionali di merci e degli investimenti. In conclusione, per tutti questi motivi e per quelli esplicitati nella relazione, che consegno, si auspica l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

ed esecuzione della Convenzione stipulata con il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e per prevenire le frodi e l'evasione fiscale, rappresenta senza dubbio uno strumento importante nel panorama delle relazioni internazionali dell'Italia. Innanzitutto, per la forma che si è scelto di adoperare, in quanto la Convenzione è stata redatta è stata redatta su uno schema fedele alle linee indicate nel modello OCSE del 1963, poi costantemente aggiornato sino al 2005. Vorrei segnalare che alla discussione in Commissione Esteri del Senato vi sono Convenzioni dello stesso tenore stipulate con Slovenia, Croazia e Bielorussia.

Comunico che il relatore ha presentato l'emendamento 1.0.300, in sostituzione dell'emendamento 1.300

Ricordo che si tratta delle sezioni che si istituiscono all'estero per i cittadini italiani, per le sole elezioni del Parlamento europeo, per coloro che non optano per votare per i rappresentanti del Paese presso il quale risiedono.

So che alcuni hanno già prospettato l'esigenza che una seduta così nutrita segua un andamento più razionale dell'usuale stillicidio di esami di singole relazioni; esse infatti spesso attengono alla medesima persona e comunque necessitano tutte di una visione complessiva sul modo in cui in questa legislatura si vuole affrontare la tematica dell'insindacabilità parlamentare. Ricordo a me stesso che oggi l'Aula è chiamata a votare su cinque proposte della Giunta concernenti l'ex senatore Iannuzzi, due proposte concernenti l'ex senatore Guzzanti, su una proposta concernente il senatore Storace e su una proposta concernente il senatore Dell'Utri. Si tratta di casi diversi e disparati che, come emergerà peraltro in modo più puntuale dall'esame di ognuno di essi, troppo spesso vengono affrontati senza tenere adeguatamente in conto le differenze che li caratterizzano. C'è una sorta di riflesso condizionato che porta in molti, troppi casi, ad esprimere un voto che dilata le prerogative parlamentari al di là della lettera e dello spirito della legge. Fuori di qui qualche tribuno parlerà di spirito di casta. Io non userò queste parole, che non condivido, così come non mi soffermerò sui costi (pure esistenti) per i bilanci pubblici che nascono da questa proliferazione del contenzioso a seguito delle frequenti sentenze di condanna sia da parte della Corte costituzionale, sia perfino da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma se vogliamo contrastare i tribuni dobbiamo imparare a fare un uso più appropriato e soprattutto meno generico e indifferente delle prerogative che abbiamo. Occorre infatti la consapevolezza di quanto delicata sia la sopravvivenza dell'immunità, come istituto esclusivamente parlamentare, evitando quell'abuso che già in passato si è rivelato foriero di una drastica delimitazione. Sarebbe controproducente un esercizio della prerogativa parlamentare che facesse venir meno le profonde ragioni per le quali i Padri costituenti apprestarono strumenti a tutela della funzione di rappresentanza democratica. Ogniqualvolta l'esercizio della prerogativa parlamentare si è sospinto al di là del limite della funzione, l'abuso del diritto ha avuto conseguenze fortemente negative

Ogni volta che votiamo a favore di insindacabilità discutibili e poco convincenti, noi rendiamo più deboli e fragili le ragioni dell'insindacabilità per quanti ne hanno titolo e diritto. Una difesa corporativa della funzione parlamentare finisce per infliggere un duro colpo oggi alla nostra credibilità e subito dopo alla efficacia delle misure che adottiamo. È quanto si è sperimentato in tema di autorizzazione a procedere con l'abuso che contraddistinse la prassi parlamentare a partire dalla fine degli anni Settanta e poi per tutti gli anni Ottanta, abuso che finì per contribuire pesantemente alla delegittimazione dell'istituto e, infine, alla sua soppressione nel 1993. È quanto si rischia di sperimentare nuovamente se si continua ad affrontare con il pilota automatico la questione dell'insindacabilità. Agire secondo stretti vincoli di maggioranza, riconoscendo sempre e comunque l'insindacabilità, significa ignorare che la Corte costituzionale ha ormai consolidato una giurisprudenza che porta inevitabilmente al capovolgimento delle decisioni parlamentari adottate nella più completa indifferenza rispetto a quella stessa giurisprudenza costituzionale, le cui linee ispiratrici sono state costantemente confermate dalla Corte. Fingere di non sapere che il vostro voto oggi, nella maggior parte dei casi in esame, non agevola la vicenda processuale di un collega, ma la ritarda soltanto significa affrontare la questione con un approccio di breve respiro, nel quale viene ad essere danneggiata la stessa funzione parlamentare che a parole si vuole difendere. Persino nel periodo asseritamente più oscuro dell'abuso dell'immunità parlamentare, nella X legislatura, ricordo che in Senato vi furono 12 concessioni su 112 richieste di autorizzazione a procedere. Invece, dall'inizio della XIV legislatura, le deliberazioni del Senato in tema di insindacabilità sono state sempre, senza eccezioni, in favore del riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare. Su 55 proposte avanzate dalla Giunta all'Assemblea del Senato, per 55 volte l'Assemblea ha deliberato nel senso dell'insindacabilità, anche quando la Giunta aveva espresso parere diverso. Si può seriamente pensare che questa sia una prassi ragionevole? Ad essere messa in discussione non è più soltanto la ragionevolezza delle singole decisioni, ma quella dell'intero assetto istituzionale della materia dell'insindacabilità e questo è un aspetto ulteriore su cui, come Presidente della Giunta, ho il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea. Ricordo a tutti che fu proprio la sentenza n. 1150 del 1988 a stabilire che la prerogativa del primo comma (la cosiddetta insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato. Questa prassi applicativa, proprio per la sua palese e manifesta irragionevolezza da un lato, e per il suo protrarsi per un ormai significativo arco temporale dall'altro, implica concretamente il rischio che la Corte costituzionale possa vedersi costretta a rivalutare le conclusioni alle quali pervenne nel 1988: è evidentemente ben difficile giustificare sul piano della ragionevolezza l'attribuzione alla Camera competente di un potere di valutare la condotta del parlamentare caso per caso, se poi questo potere viene esercitato in concreto valutando sempre tutti i casi nello stesso modo e con il medesimo esito. Questo è il punto.

Signora Presidente, concordo pienamente con quanto il presidente Follini ha detto ora e non ho molto da aggiungere al problema che è stato posto. Indipendentemente dell'opinione che ciascuno di noi può avere sul rapporto tra istituzioni, tra poteri dello Stato,

una giurisprudenza della Corte costituzionale, ormai costante dal 2000, che in tema di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione sull'insindacabilità lega le condotte che i parlamentari parlamentari tengono al di fuori dell'Aula parlamentare alla loro attività interna al Senato o alla Camera. In altri termini, se un senatore, in un comizio, in una trasmissione televisiva o in qualsiasi occasione pubblica, occasione pubblica, formula un'opinione che possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale, di per sé la qualifica di parlamentare non fa scattare automaticamente vi è la necessità che la dichiarazione o il comportamento siano collegati in maniera specifica ad un'attività parlamentare: un atto ispettivo, un'iniziativa legislativa o quant'altro. da nove anni a questa parte, per nove anni la Corte costituzionale ha dato torto al Parlamento ogni qualvolta questo abbia dichiarato l'insindacabilità di un parlamentare al di fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla Corte, oneri aggiuntivi a carico del Parlamento e ovviamente un calo del livello della credibilità delle decisioni che noi assumiamo.

di un conflitto tra diverse opinioni politiche e parlamentari. Il tema è molto più concreto e pragmatico, se così vogliamo dire, di quanto non appaia:

Abbiamo, dicevo, due strade: o modifichiamo l'articolo 68 e precisiamo che l'insindacabilità riguarda anche, in maniera generale, l'attività parlamentare *extra moenia*; oppure, fin quando questo non avviene, dobbiamo attenerci alle sentenze della Corte costituzionale.

sospensiva di alcune delle relazioni iscritte all'ordine del giorno punta sostanzialmente a non esaminare tutti quei casi rispetto ai quali è certo,

abbiano la copertura della insindacabilità perché rientrano nell'ambito delle previsioni costituzionali, così come interpretate dalla Corte. Questo è il senso della mia proposta e mi auguro che i colleghi ne possano far tesoro.

del senatore D'Alia affronta un problema di una estrema delicatezza. È vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale nel corso di questi anni è stata particolarmente dura nei confronti delle decisioni delle Camere: c'è una giurisprudenza costante della Corte costituzionale proprio sul punto dell'articolo 68.

del 2003, che riguarda l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, all'articolo 3 individua le attività del parlamentare coperte dall'articolo 68 della Costituzione. In detto articolo 3 si fa riferimento non soltanto alle attività tipiche del parlamentare, quali le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze, ma si dice che l'articolo 68 si applica per ogni altro atto parlamentare e per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori del Parlamento. Questa è la legge.

con la sentenza n. 120 del 2004, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3,

con l'ordinanza del 23 gennaio 2006, n. 37, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale e manifestamente infondata la questione in riferimento all'articolo 3, comma 1. l'articolo 3, comma 1, viene dichiarato legittimamente e costituzionalmente orientato, tant'è vero che la Corte

Non mi convince la decisione di sospendere tutto e aspettare che qualcosa cambi, sperando che nel giro di un anno la Corte costituzionale possa orientarsi e orientarci un po' meglio: non è una decisione che riesco a comprendere. Può il Parlamento fermarsi di fronte a delle richieste? Ritengo che la sospensione di un anno in attesa non di un atto che è già all'ordine del giorno, ma di un qualsiasi evento che potrebbe forse accadere sia del tutto improponibile. Pertanto, sono dell'opinione che il Parlamento debba continuare ad applicare le sue prerogative nel rispetto delle leggi nel rispetto delle leggi attualmente in vigore e poi sarà la Corte costituzionale, quando sarà investita, a dire se facciamo bene o male. Signora Presidente, do atto al presidente Follini di aver posto un tema serio, sia nelle argomentazioni sia nei toni; di fronte a questa riflessione le nostre orecchie non sono insensibili. Penso però che tutti dovremmo riconoscere, indipendentemente da qual è il nostro pensiero, che in questa materia si è rotto un equilibrio originario. Richiamiamo l'equilibrio costituzionale ogni qualvolta ciò serva anche a scopi politici immediati e spesso a sproposito. In questa materia non dobbiamo dimenticare che la Costituzione nell'equilibrio di *checks and balances* previsto originariamente per regolare i rapporti tra la politica e la giustizia prevedeva l'istituto dell'immunità parlamentare. È caduto quell' istituto ed il sistema ha perso il suo equilibrio. La mancanza di un equilibrio si può ammettere, indipendentemente da ciò che si pensa su quella riforma dell'originario impianto costituzionale. In questo senso, la cosa è anche certificata. Si è richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale giustamente, ma una considerazione di quella giurisprudenza mette in evidenza che essa non ci dà delle indicazioni univoche. Se si fa un esame attento delle sentenze si scorgono non poche contraddizioni. Possiamo cercare di ripristinare un nuovo equilibrio. Possiamo farlo fino al punto che ci indicava il collega D'Alia di rimettere in discussione l'articolo 68 della Costituzione, e lo possiamo fare rivedendo la giurisdizione domestica. Ma questo è il tema che dovremmo affrontare nelle sedi proprie, iniziando da quell'esame di revisione dei Regolamenti che dall'inizio della legislatura abbiamo assunto come impegno, ma che fino ad ora non siamo riusciti a portare avanti.

ponendo questo blocco sulle spalle delle persone che per caso sono rimaste coinvolte in questo determinato momento. Questo è il motivo per cui, nel momento stesso in cui chiediamo all'Assemblea di andare davanti e assumersi le proprie responsabilità, non chiudiamo assolutamente la porta ad una riflessione che anche noi riteniamo necessaria. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una breve considerazione è doverosa dopo l'intervento del presidente Follini, che ricordo riveste un ruolo di garanzia. Non si è espresso in Aula, almeno così credo, come *leader* politico di opposizione, ma come il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il massimo organo di garanzia per questo ramo del Parlamento. Ho sentito espressioni però che, al di là dei toni usati, sono molto forti. presidente Follini ha parlato di difesa corporativa, di scudo di cartone, di pilota automatico. Poiché io, assieme a tanti altri colleghi, faccio parte di questa Giunta, non ritengo davvero di poter accettare queste affermazioni così pesanti; riteniamo infatti di aver svolto e di svolgere quotidianamente un lavoro importante, che tiene conto della giurisprudenza parlamentare, colleghi. Non dimentichiamoci che esiste una giurisprudenza parlamentare. Dal 1947 l'articolo 68 è stato applicato tantissime volte dalle varie Giunte che si sono susseguite e si è formata una giurisprudenza parlamentare che per me, senatore di questa Repubblica, vale di più della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha mutato nel tempo i suoi orientamenti, perché la Corte costituzionale non vive in un mondo astratto ma in un mondo dinamico che sta cambiando. È la stessa Corte che ci ha detto nel 2007 che occorre adeguare la garanzia dell'insindacabilità alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento dell'attività politica. Oggi l'attività politica è estremamente dinamica, con caratteristiche particolari. Ecco la difficoltà per la Giunta di affrontare anche questo tema della insindacabilità a fronte di una attività completamente mutata nel tempo. Ma il nostro parametro di riferimento è sempre, e deve essere sempre, la giurisprudenza parlamentare. Quindi, sinceramente respingiamo al mittente le accuse di difesa corporativa: non operiamo come difensori della corporazione e della casta, semplicemente applichiamo una prerogativa funzionale che difende una funzione parlamentare importante per il nostro Paese. Presidente, voglio affrontare la questione che è stata così serenamente ed anche opportunamente sollevata dal senatore Follini e poi ripresa dal senatore Quagliariello, in quanto è delicatissima. Ha ragione il senatore Quagliariello: stiamo ragionando di quel delicatissimo equilibrio di *checks and balances* che, in un sistema come il nostro, garantisce l'impianto costituzionale e garantisce anche contro squilibri che questo sistema (non è un inciso polemico, lasciatemelo dire) ha di recente conosciuto con l'approvazione del cosiddetto lodo Alfano, fonte peraltro neanche credo sia opportuno tornare sulle ragioni del presidente Follini e fare un passo indietro, alla stagione nella quale il ricorso alla alla consultazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere nei due rami del Parlamento era frequentissimo perché, come tutti ricordano, fu una stagione di molte indagini che riguardavano appartenenti alla Camera e al Senato.

istintivamente ed emotivamente contro il potere; si assisteva ad episodi che apparivano inspiegabili: si aggredivano uomini politici che non si erano mai conosciuti, con cui non si aveva mai avuto niente a che fare, perché in realtà erano i rappresentanti di un potere istituzionale avvertito come sordo, lontano, ingiusto e disattento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle cittadine.

necessario da difendere: quell'esercizio libero della funzione parlamentare, cara ai Costituenti e preziosa per la Costituzione, in un Paese che veniva da anni di persecuzioni politiche e di limitazione dei poteri del Parlamento e della libertà della funzione parlamentare per i tanti che si erano schierati contro il Governo Mussolini. strumento delicatissimo che, come ci insegna il professor Quagliariello, andava usato nei limiti del proprio rigoroso campo di esercizio, perché se fosse esondato - come esondò un uso arbitrario e tutto difensivo di una corporazione, era ovvio che avrebbe perso non solo la sua nobiltà ma proprio la sua funzione principale in un sistema democratico: quella di difendere

ma paradossalmente ci ha richiamato, con maggiore rigore di quanto non facessero l'articolo 68, la giurisprudenza parlamentare e la stessa giurisprudenza costituzionale e di merito, ad un uso responsabilità. Perché ogni volta che una Camera di appartenenza decide sulla non concessione decide in realtà una sorta di conflitto di attribuzione, stabilendo a chi tocca il potere, e quindi quella funzione di bilanciamento - già così presente nella Costituzione del 1948 - è diventata ancora più pregnante perché ogni Camera definisce il proprio ambito sostanziale di giurisdizione e di attribuzione tutte le volte in cui, con questo articolo 68, viene a decidere.

invece che il richiamo fatto dal presidente Follini sia da questo punto di vista prezioso. In qualche modo, oggi, la responsabilità che grava sulle Aule di Montecitorio e di Palazzo Madama ogniqualvolta decidono su un'autorizzazione a procedere è ancora più più gravosa di quanto non fosse con l'articolo 68. Quindi, l'invito ad un uso rigorosissimo del nostro voto credo sia

la suggestione del bel tempo antico e la tentazione di tornare ad un regime dell'articolo 68 che fu modificato all'unanimità - voglio ricordarlo - nel 1993.

l'articolo 68 fu modificato - per ben dieci anni si dibatté in Parlamento alla ricerca di una soluzione che potesse essere coerente, concretamente coerente, con quelle che erano le esigenze della tutela del Parlamento.

che il senatore Follini ha rappresentato all'Aula e l'*excursus* storico che la senatrice Finocchiaro ha poc'anzi proposto. La legge - quella che va applicata, la legge di attuazione e l'analisi delle condotte del parlamentare - prevede che il parlamentare possa divulgare, criticare e denunziare politicamente. Il mandato che viene conferito non può essere ingabbiato nella tipicizzazione di alcune condotte. Tutto ciò che io critico, il mio dissenso a volte esasperato, lo debbo rassegnare all'interrogazione, alla mozione, all'interpellanza oppure alla discussione in quest'Aula? Di ciò si è reso interprete il legislatore del 2003 e questa legge e questa legge fece. Se questa è la legge, non vedo quali Regolamenti interni del Senato possano modificare questo assetto, che è puntuale, rigoroso e preciso.

che viene proposto all'Aula, credo ricomprenda tutte le critiche, gli apprezzamenti e le contrapposizioni che hanno caratterizzato il dibattito nel corso dei lavori della Giunta. Quindi, Presidente, se le condotte si rifanno all'esigenza divulgativa della propria attività politica o alla critica, ebbene, la politica ormai non è soltanto quella che si svolge all'interno delle Aule parlamentari e con gli atti tipici, come tutti sappiamo. Ho poca dimestichezza con il *web* e con Internet, poiché appartengo forse a un'altra generazione, quella della penna rossa e della penna blu. Mio malgrado, non sono riuscito a cogliere appieno questa esigenza di modernità, ma il dato è incontrovertibile: la politica ormai è varia e i meccanismi attraverso i quali il pensiero politico dell'eletto giungono alle aree vaste della società

a mio avviso, interpretazioni di sorta. Queste condotte così caratterizzate, fino alla denunzia politica, sono incensurabili e rientrano nelle previsioni dell'articolo 68.

vorrei intervenire sulle modalità di voto. Ho raccolto prima - e credo che lei me lo confermi - l'intenzione della Presidenza di sottoporre all'Aula la questione mediante voto palese.

la richiesta di voto segreto. Come tutti sappiamo (è scritto anche nell'edizione del Regolamento che è affidata a questa legislatura), l'articolo 113 del nostro Regolamento, sulle questioni che attengono alle persone o alle libertà fondamentali stabilite dalla nostra Costituzione agli articoli 13 e seguenti, prevede la possibilità del voto segreto.

distinse e stabilì che per l'autorizzazione all'arresto, trattandosi di libertà personali, si usava il voto segreto, mentre per le autorizzazioni a procedere (che oggi, come sappiamo, non esistono più),

Noi riteniamo che la questione che attiene alla insindacabilità delle opinioni dei parlamentari riguardi la libertà di espressione del parlamentare

che parlava di autorizzazione a procedere. Quelle che abbiamo oggi davanti non sono autorizzazioni a procedere, bensì valutazioni sull'insindacabilità dell'opinione dei senatori che

dalla nostra Costituzione all'articolo 21, della libertà di espressione. Ripeto: una libertà specificata e sottolineata con maggiore spessore perché legata alla funzione parlamentare, ma sempre

di vedere valutata dall'Aula, nel pieno della sua libertà, la tutela della funzione parlamentare, ma c'è anche un aspetto della questione che attiene alla libertà di espressione dello stesso parlamentare e del cittadino. Le chiedo quindi la possibilità di votare al voto segreto Onorevoli colleghi, in merito all'ammissibilità di richieste di votazione a scrutinio segreto sulle insindacabilità parlamentari, la Presidenza non può che tener conto del parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993. In forza di quel parere fu innanzitutto escluso che le autorizzazioni a procedere, a quel tempo previste dalla Costituzione, potessero rientrare nel novero delle votazioni concernenti persone, costituendo le stesse espressione di una prerogativa dell'organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri organi dello Stato. Tale parere, da allora, è stato costantemente ritenuto applicabile anche alle questioni di insindacabilità. Il parere stabilì inoltre che in applicazione dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti l'arresto, la perquisizione personale e domiciliare, nonché altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni citate ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione. Infine, appare di tutta evidenza che le delibere di insindacabilità hanno un riflesso soltanto mediato sull'articolo 21 della Costituzione e quindi non può che discenderne l'inammissibilità della richiesta di votazione a scrutinio segreto motivata dal riferimento a tale disposizione costituzionale.

*(PD)*. Signora Presidente, mi rifaccio proprio alle sue ultime parole e ad un'espressione che è contenuta nel parere che è stato dato nella valutazione della Presidenza in ordine alla nostra richiesta di procedere con voto segreto.

nel senso che si tratta, sia tecnicamente che giuridicamente, ma anche sostanzialmente, di una valutazione che è stata espressa esclusivamente dalla Giunta

il quale cita una serie di articoli della Costituzione non in maniera casuale, ma in modo molto specifico e dettagliato e con un contenuto sostanziale. perché oltre a fare riferimento alla norma ricordata dal collega Sanna, quella dell'articolo 21 della Costituzione, il nostro Regolamento cita altre norme costituzionali

che è stata senatore e nostro collega in quest'Aula. Si tratta, quindi, di un insieme di questioni attinenti anche ad altre norme della nostra Carta costituzionale. Ne cito alcune rapidamente: innanzitutto, l'articolo 13 sulla libertà personale inviolabile; inviolabile; l'articolo 21, che è già stato citato, ma anche gli articoli 24 e 27 sulla responsabilità penale, ancora sulla libertà delle persone e sul collegamento del fatto rispetto alla previsione normativa penalistica.

il quale, per definizione, ha a che fare con responsabilità penale e con responsabilità delle persone, con tutte le conseguenze chiaramente e facilmente intuibili da parte di tutti.

Per il momento, la Presidenza non può che ribadire l'inammissibilità del voto segreto.

La prima questione è la seguente: è evidente che ci troviamo di fronte ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge che disciplina la materia. Vi è però un dato reale del quale dobbiamo purtroppo prendere atto, perché non rendiamo neanche un buon servizio ai nostri colleghi che si trovano di fronte o esposti ad un'iniziativa giudiziaria. Dal 2000 ad oggi, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, in alcuni casi il Parlamento è risultato soccombente. e ci assumiamo la responsabilità d'intervenire legislativamente anche a livello costituzionale, oppure dobbiamo prendere atto di ciò. L'unica cosa che non possiamo fare è continuare a produrre deliberazioni sistematicamente censurate dalla Corte, perché questo non è né serio né corretto

che riguarda il lavoro futuro della stessa Giunta, perché è evidente che o ci atteniamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale - e poi l'Aula legittimamente smentisce

Signora Presidente, avrei preso anch'io molto volentieri la parola sull'importante relazione del presidente Follini e sul dibattito che

Presidente, lei ha fatto riferimento ad una decisione della Giunta del Regolamento del 1993. Dopo il 1993 molte cose sono cambiate, come abbiamo sentito negli interventi che si sono succeduti. Le chiedo, per cortesia, di voler valutare la possibilità di sospendere l'esame delle questioni per le quali l'Aula è stata oggi chiamata a discutere,

sono molto lontani e appaiono superati da tutta la normativa successiva. Penso che oggi siamo stati chiamati a trattare questioni che - come ha ricordato il presidente Follini la Giunta si trascina da un bel po' di tempo. Se aspettiamo ancora qualche ora o qualche giorno per affrontarli, avendo sciolto il tema delle modalità di voto, credo che faremmo bene al Senato. *(Applausi dal

mi sembra che ci sia stata una discussione importante in quest'Aula. Però, colleghi, non scherziamo. Non apriamo un dibattito sulle decisioni della Presidenza. Né possiamo ritenere che un Regolamento è valido fino a un certo punto, dopodiché lo si mette in discussione. Sono stato il primo a dire che la questione investe anche la modifica del Regolamento, soprattutto in relazione alla alla giurisdizione interna alla quale ha fatto riferimento il presidente Follini. Ma finché il Regolamento è questo, per quello che ha dichiarato il Presidente sono queste le regole del gioco.

è intervenuto sollevando una questione che attiene alle modalità del voto, cioè al voto segreto, e ha detto che la materia è stata regolata dal Senato sulla base di una opzione scelta molti anni fa,

neanche per decisioni assunte dalla Giunta in epoca molto più prossima rispetto a quella cui ha fatto riferimento il senatore Casson. Qual è il problema perché l'Aula di fronte ad una questione sollevata non ritenga di poter investire la Giunta per il Regolamento?

senatore Francesco Storace, chiamato dalla magistratura ordinaria a rispondere in un procedimento penale che pende presso il tribunale di Roma

tra le cose che fanno parte della sua attività parlamentare tipica (le interrogazioni, gli interventi in Aula, le proposte di legge e così via), nulla c'entravano queste che, secondo un'ipotesi accusatoria che non spetta a noi valutare, vengono ritenute dalla magistratura come fattispecie ricadenti nell'articolo 278 del codice penale. Quindi, a noi non spetta oggi giudicare l'ex senatore Storace riguardo ad accuse gravi rispetto alle quali il Presidente della Repubblica non può difendersi, perché non si è mai visto un Presidente della Repubblica che quereli un cittadino o un o un parlamentare o l'espressione di una qualsiasi opinione nei suoi confronti. Non si è mai visto perché, accanto alla sua irresponsabilità costituzionale c'è questa norma che è l'unica tutela che ha il Presidente della Repubblica. È una tutela che gli viene garantita dall'ordinamento. Pertanto,o decidiamo di abrogare l'articolo 278 del codice penale oppure dobbiamo valutarlo alla stregua di tutte le altre opinioni che i parlamentari esprimono. Non c'è alcuna relazione, alcun nesso funzionale tra l'attività

reinterpretata dalla Corte costituzionale che invece ha ristretto in maniera puntuale a reati tipici e all'attività parlamentare questo tipo di di tutela, di garanzia e di immunità. Noi non rientriamo nell'ambito di questa tutela e del perimetro di questa immunità. Stiamo andando un'altra volta incontro ad un giudizio di conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale che molto probabilmente perderemo. Noi non vogliamo essere quelli che di fronte a tale prospettiva oggi sono stati zitti.

parlamentari è stata già stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ravvisando l'insussistenza dei presupposti procedurali per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del senatore Dell'Utri, ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Chiedo al relatore, senatore D'Alia, se intende intervenire.

Si tratta del caso, che ci viene sottoposto dal tribunale di Palermo, di richiesta di poter utilizzare le intercettazioni indirette del senatore Marcello Dell'Utri.

merito della rilevanza di queste intercettazioni (posto che non è la Giunta o il Senato che devono valutare la rilevanza),

Tuttavia, quella che dobbiamo applicare è una legge che in termini di lettura di un procedimento penale ordinario attribuisce al giudice delle indagini preliminari

nel sottoporci questa richiesta. È questo il senso del voto a favore delle conclusioni della Giunta. Signor Presidente, in questa fattispecie la Giunta propone la restituzione degli atti al giudice richiedente, in quanto si assume, da parte della maggioranza della Giunta, che l'organo deputato a chiedere alla Camera l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 sia il giudice del fatto e non il giudice dell'udienza preliminare. Vorrei far presente che in materia di intercettazioni esiste un giudice delle intercettazioni, che è il giudice delle indagini preliminari, cioè il giudice che autorizza le intercettazioni o meno. Tutto ciò che riguarda le intercettazioni, ossia la loro utilizzazione fino al punto della loro distruzione, distruzione, che può essere richiesta anche quando il processo sia nei gradi successivi di giudizio, deve essere deciso sempre dal giudice che adottò il provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni. È una procedura, quindi, estremamente garantita. La magistratura palermitana intende utilizzare in diverso procedimento le intercettazioni che riguardano il senatore Dell'Utri. Si dice nella proposta della Giunta che questa richiesta deve poter essere articolata dalla corte d'appello. Sennonché, per poter la corte d'appello pronunziarsi sull'utilizzazione, i documenti costituenti l'intercettazione devono essere depositati il giudice di Palermo ritiene che il deposito stesso della documentazione al giudice del fatto costituisca utilizzazione, sicché per poterutilizzare questa documentazione deve avviare la procedura di autorizzazione da parte delle Camere. È una procedura garantita, che si vuole applicare. Dire che deve essere il giudice del fatto a formulare questa richiesta è qualcosa che va contro il nostro sistema: il giudice delle intercettazioni è il giudice delle Questo è previsto espressamente dall'articolo 270 del nostro codice di procedura penale e non possiamo noi imporre ad un altro organo di fare qualcosa che il sistema non prevede. C'è un giudice delle intercettazioni, quindi dobbiamo esaminare se sia garantista la procedura seguita dall'autorità giudiziaria di Palermo. Non possiamo dire che intanto chi chiede l'autorizzazione depositi gli atti al giudice del fatto e poi sarà il giudice del fatto a decidere, perché già il momento del deposito dei documenti nel fascicolo del giudice che deve decidere è utilizzazione. Si chiede quindi di essere autorizzati a questo deposito e la richiesta non può se non farsi da parte del giudice che ha disposto le intercettazioni. Non ha senso assumere che il giudice che dispose le intercettazioni e che oggi fa la richiesta di autorizzazione sia un giudice che non conosca: non vuol dire nulla, questo. Vi è un giudice già individuato dal nostro sistema, il giudice delle intercettazioni; non possiamo non possiamo spostare la competenza. La conferma di questo è proprio prevista dal nostro sistema nel momento in cui, a proposito delle intercettazioni che possono farsi per la ricerca dei latitanti, introduce l'unica eccezione del sistema stesso, ossia quando stabilisce che per la ricerca di latitanti - questa ipotesi è anche analizzata nel corso della relazione

prevista dall'articolo 295, comma 3-*ter*. Essendo questa l'unica eccezione, per il resto si applica la procedura normale. Ora, io ritengo che restituire gli atti all'autorità giudiziaria per dire che debba provenire una delibazione e una richiesta da parte della corte d'appello, ossia del giudice del fatto, sia qualcosa giuridicamente errato. Applichiamo il codice così come disciplina la materia; non esponiamo il Parlamento ad una ad una valutazione molto censurabile dal punto di vista tecnico. Ecco perché riteniamo che correttamente e in forma garantita la proposta a noi pervenga da parte del giudice che dispose le intercettazioni, l'unico competente a valutare tutto tutto quello che riguarda utilizzazione e distruzione, anche a distanza di anni, di quelle intercettazioni autorizzate. Quindi, non riteniamo che possa essere accolta la proposta della Giunta con cui si chiede che sia la corte d'appello a formulare una richiesta, il che presuppone già un'utilizzazione di atti che invece, ai sensi della legge n. 140 del 2003, devono essere vagliati dalla Camera di appartenenza del parlamentare. Voteremo pertanto contro la proposta della Giunta.

(correttamente, riteniamo noi), al giudice del fatto, cioè alla corte d'appello, la quale è l'unica che può valutare la rilevanza ai fini della utilizzazione di questa intercettazione che, peraltro, nella fase del giudizio di primo grado, non sembra essere stata né richiesta né utilizzata. La seconda considerazione è che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, che fa esplicito riferimento, come dice il collega Li Gotti, al giudice per le indagini preliminari nella individuazione dell'organo giurisdizionale competente a richiedere l'autorizzazione, non è e non può ritenersi esaustivo delle ipotesi; infatti, la formulazione che il legislatore ha utilizzato si spiega supponendo che lo stesso abbia inteso considerare espressamente la situazione di fatto più frequente, ma sarebbe eccessivo desumere da ciò che la richiesta di autorizzazione possa essere formulata solo dal giudice per le indagini preliminari. Al riguardo, faccio un esempio di ordine testuale. Il vigente codice di procedura penale prevede che le intercettazioni processualmente utilizzabili siano autorizzate (o convalidate) dal giudice per le indagini preliminari in via ordinaria, ma non esclusiva, posto che l'articolo 295 del codice, nel consentire il ricorso alle intercettazioni al fine di agevolare, ad esempio, la ricerca del latitante, prevede - mediante il rinvio agli articoli 268, 269 e 270 del codice medesimo - che le stesse siano utilizzabili anche ai fini probatori, stabilendo inoltre che tali intercettazioni possano essere disposte dal giudice o dal pubblico ministero (e precisando ulteriormente che nei giudizi davanti alla corte d'assise in luogo del giudice provvede il presidente della corte), senza quindi alcun esclusivo riferimento alla figura del giudice per le indagini preliminari. Da ciò deriva che la tesi fatta propria dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo porterebbe alla conclusione che, nelle ipotesi di intercettazioni disposte per la ricerca del latitante da un giudice diverso, in una fase del procedimento successiva alle indagini preliminari, delle stesse non si potrebbe mai richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione perché mancherebbe il soggetto legittimato a farlo, con conseguente irrimediabile (e ingiustificabile) pregiudizio per le finalità di accertamento del procedimento penale.

che risultano incompatibili con la lettera della stessa legge n. 140 del 2003. Questa, infatti, prevede il giudizio sulla necessità di utilizzare l'intercettazione come presupposto necessario della formulazione della richiesta di autorizzazione alla Camera competente (si veda in tal senso il comma 2 del citato articolo 6). di elementi probatori, l'unico soggetto legittimato in base al codice a poter fare tale valutazione è il giudice che ha cognizione della causa, non un giudice diverso ed estraneo. Diciamo che è stata utilizzata

con l'autorità giudiziaria, tende a far sì che si segua il procedimento corretto, a garanzia del diritto del contraddittorio, del diritto di difesa e della genuinità della prova. Queste le ragioni che ci hanno portato a tale conclusione, pressoché unanime, in Giunta.

Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

e che hanno a che vedere con dichiarazioni da lui rese a mezzo stampa nell'esercizio della sua professione. In sostanza, attraverso articoli sul quotidiano «il Giornale», il senatore ha sostenuto delle tesi nei confronti dei diversi querelanti e, a procedimento avviato, il difensore ha chiesto l'insindacabilità ai sensi della normativa vigente. Noi su tutti questi provvedimenti voteremo

la Giunta si è espressa in maniera diversa rispetto alla mia opinione, alla mia proposta, e quindi è stato nominato un altro relatore, il collega Mazzatorta. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto: stiamo affrontando, infatti, nel dibattito un po' generale che ha visto quest'Aula riflettere sulle questioni di insindacabilità un aspetto molto particolare. In sostanza, tutta la difesa che viene fatta propria dal relatore di maggioranza si basa su un elemento, cioè l'impossibilità di scindere

cui non è possibile distinguere quando un collega opera come senatore (e quindi le sue dichiarazioni hanno una stretta attinenza con la sua attività di senatore, con gli atti che compie in questa sede, con le sue proposte di legge, le sue interrogazioni, le sue dichiarazioni in quest'Aula)

che esercitano una professione, siano essi avvocati o medici o quant'altro), noi non possiamo pensare di introdurre con il nostro voto una nuova fattispecie protetta costituzionalmente che prevede

nella lunga audizione che abbiamo tenuto, molto esplicitamente e con una sincerità che è stata apprezzata da tutti i colleghi, ma che ci motiva nel nostro voto contrario, egli ha sostenuto

perché era diventato senatore in quanto giornalista. Questo è un ragionamento che potrebbe fare qualsiasi stimato collega di altre professioni

Ciò è grave, per cui invito a una riflessione serena su questo punto, che è diverso da tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima e che va nella specificità di questi casi.

come si è visto nella votazione precedente e le altre volte. Vorremmo, per la dignità di questa nostra istituzione, che tutti i colleghi cercassero di fare un simile sforzo. Ogni caso va guardato per quello che è. è. Se non vogliamo trovare da parte della Corte costituzionale un atteggiamento pregiudizievole, dobbiamo essere sempre in grado di motivare nel merito ogni provvedimento, come ho modestamente cercato di fare.

Signor Presidente, mi rimetto alla

giustificata dal fatto che ero relatrice del provvedimento, ma poi il voto della Giunta ha modificato l'orientamento da me proposto. Alle considerazioni che ho svolto precedentemente, invitando tutti ad

l'ora e la stanchezza, però stiamo discutendo di temi estremamente delicati, che riguardano nostri ex colleghi, e seguendo gli interventi di relatori di maggioranza e di minoranza. Tra l'altro, ho preso atto che questa mattina c'è stato un ampio dibattito su argomenti che

che comprende ma va oltre - dalle questioni di ordine generale discusse precedentemente e che richiederebbero un ripensamento da parte della Giunta (come peraltro sollecitato dai due Presidenti delle Camere), ripensamento che ci accingeremo a fare quando sarà possibile. Noi qui rigettiamo la richiesta della magistratura e diciamo che sono insindacabili

Inoltre, aggiungo alle considerazioni già fatte altre due. *In primis*, la legge in vigore - che non ha certo valore costituzionale, ma è pur sempre una legge in vigore - prevede che, se venisse eletto un direttore di giornale,

Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro gli esiti della Giunta. Noi partiamo da un principio, un principio, quello di un'uguaglianza dei cittadini che non può essere forzata soltanto per i parlamentari. Quindi, noi riteniamo che sia giusto che i parlamentari, come gli altri cittadini, siano oggetto di giudizio nelle sedi opportune possano difendersi ovvero prendere un altro tipo di iniziative per difendere le proprie opinioni, i propri orientamenti e perseguire coloro i quali, eventualmente, abbiano offeso

parlamentari è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo alla relatrice, senatrice Adamo, se intende intervenire.

in entrambi i casi, valutando gli atti e le dichiarazioni rese in Giunta, ero arrivato alla conclusione di un voto favorevole in un caso e contrario nell'altro.

prima puntualmente il Presidente della Giunta - a logiche che valutino nel merito. Ognuno di noi, indipendentemente dall'appartenenza politica, deve tenere questo comportamento, nella Giunta e in quest'Aula, quando si affrontano questioni di questo tipo.

non consente un'automatica estensione delle prerogative e delle guarentigie assicurate dall'articolo 68 della Costituzione. giustifica l'intervento che il senatore Iannuzzi fece all'epoca proprio perché collegato anche alla sua attività di parlamentare, essendo stato il senatore Iannuzzi primo primo firmatario della proposta di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, atto comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2004 e ricordo che, nella relazione di accompagnamento, erano stati menzionati vari episodi sintomatici di un uso se non distorto quanto meno dubbio della funzione e del ruolo del collaboratore di giustizia. È pertanto questo un atto tipicamente parlamentare. Quindi, quand'anche si accedesse alla tesi più restrittiva e all'interpretazione condotta dalla Corte costituzionale sulla latitudine del mandato del parlamentare, sicuramente le riflessioni e l'azione di denunzia politica fatta dal senatore Iannuzzi con quell'articolo sono certamente riferibili ad un atto parlamentare di cui egli

viene argomentato con il richiamo all'articolo 3, comma 4, della legge sulla libertà di stampa. Mi permetto di osservare che questa disposizione riguarda specificamente la funzione di responsabilità che è riconosciuta al direttore responsabile di un quotidiano e all'obbligo che egli ha di rassegnare le dimissioni qualora rivesta mandato parlamentare. Siamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità completamente diversa, perché è quella che attiene alla vigilanza su quanto viene pubblicato nel giornale, quindi alla complessità non solo degli articoli ma perfino delle inserzioni, della pubblicità e di quant'altro. Pertanto, abbiamo di fronte una situazione completamente diversa del parlamentare che attraverso un quotidiano, quindi attraverso un articolo, svolge la sua funzione di denunzia politica, così come è avvenuto in questo caso, e in modo assolutamente conforme alla norma che disciplina la funzione del parlamentare, così come è stato ricordato anche nel dibattito che ha preceduto le votazioni. dalla Giunta e, comunque, non aderendo alle conclusioni rassegnate nella relazione dalla Giunta stessa, riteniamo che la vicenda e le espressioni rese dall'allora senatore Iannuzzi siano sicuramente riconducibili alla situazione di non sindacabilità *ex* articolo 68, primo

sulla questione complessa dell'estensione, interpretazione ed applicazione dell'articolo 68, mi muovo in un'ottica estremamente precisa. Nel caso che stiamo esaminando non giudichiamo una richiesta che riguarda delle opinioni espresse: ciò che è materia del processo e per cui si chiede alla Camera dei deputati di valutare la sindacabilità o meno sono fatti, non opinioni. Nell'articolo in questione l'ex senatore Iannuzzi espresse delle opinioni sulla base di un'affermazione in fatto. L'opinione era corretta rispetto al fatto da lui riferito, quindi opinione corretta, sennonché era il fatto sbagliato, ossia era un fatto inventato. Sulla base di questo, non ritengo che si possa tutelare l'opinione quando quest'ultima contenga l'affermazione di un fatto che è contro verità, perché diversamente, se si costruisce un fatto falso, poi tutte le opinioni sono legittime. Allora, in una vicenda del genere, non ritengo che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, che riguarda l'attività dei parlamentari negli atti tipici e negli atti atipici, possa riguardare anche l'affermazione di fatti specifici contro verità. il mio voto sarà in conformità alle deliberazioni della Giunta

richiamare ancora una volta che se la legge che lo stesso senatore Sarro ha citato chiede addirittura le dimissioni del direttore per un giornalista che è quello che esprime

il fatto di aver chiesto la formazione di una Commissione d'indagine, non su questi fatti ma in generale su una casistica, è esattamente uno dei punti che è contestato in tutte le sentenze della Corte costituzionale, per tornare al problema come ci è stato posto all'inizio. ovvio che qualsiasi cosa può essere attinente al lavoro di un parlamentare, in questo caso una Commissione d'indagine sull'uso dei pentiti, ma su questa vicenda specifica il senatore cosa ha fatto? Nulla come senatore.

Colleghi, vogliamo far concludere la senatrice Adamo, per cortesia? La seduta terminerà alle ore 13,00 e tra l'altro verrà

nuova finestra"). Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha definito modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori per la settimana successiva alla prossima, fino al 5 marzo. Nella seduta pomeridiana di martedì 24 febbraio - dalle ore 16 alle ore 21 - è anticipata la discussione delle mozioni sulla crisi dei mercati finanziari. Per tale dibattito ciascun Gruppo avrà a disposizione 30 minuti, comprensivi di illustrazione, interventi in discussione generale e dichiarazioni di voto. Dopo il voto delle mozioni sarà esaminato il disegno di legge collegato su produttività lavoro pubblico, con l'auspicio

in luogo del sindacato ispettivo), sarà discusso il disegno di legge collegato su semplificazione e processo civile. Per i due disegni di legge collegati si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nelle sedute della settimana 3-5 marzo, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato sul processo civile, sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sulle quote latte. Anche per questo provvedimento i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. Nella seduta antimeridiana di giovedì 5 marzo, alle ore 11, sarà avviata la discussione dei disegni di legge sul testamento biologico con la relazione del relatore, il voto di possibili questioni incidentali ed eventualmente qualche intervento in discussione generale.